che, unitamente ad altri senatori, richiamano l'attenzione sulla ventilata chiusura di una serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni sul territorio nazionale, tra le quali quelle di Pordenone, Gorizia, Modena e Foggia. le interrogazioni dei senatori Albano e Vaccari sono state presentate diverso tempo fa (risalgono al 2014), ma ritengo che la risposta possa ancora essere di loro interesse, in quanto il tema trattato nei rispettivi atti mantiene tuttora caratteri di stretta attualità, dopo essere rimasto aperto per tutti questi anni in forza di sopravvenienze normative - di cui parlerò tra un attimo - che ne hanno condizionato l'evoluzione. La questione della chiusura di alcune sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni, è legata, al pari della proposta di soppressione di altri uffici di polizia sul territorio nazionale, all'attuazione di un piano di razionalizzazione sottoposto al parere delle autorità provinciali di pubblica sicurezza nei primi mesi del 2014. Il piano è ancora in attesa di definizione, anche a causa dell'approvazione della legge n. 124 del 2015, con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare importanti misure di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Per quanto attiene in particolare al riordino del sistema della pubblica sicurezza, legislatore ha chiarito che il nuovo assetto organizzativo dovrà essere volto a evitare duplicazioni e sovrapposizioni dispersive nell'esercizio delle funzioni di polizia, nonché favorire la gestione associata dei servizi strumentali in adesione ai principi di efficienza della spesa pubblica. Tali principi sono stati recepiti nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, con cui è stato stabilito che la razionalizzazione della dislocazione delle forze di polizia sul territorio sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei Comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, fatte salve specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Per giungere alla compiuta definizione di tale disegno di valenza strategica, sono stati istituiti, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, appositi gruppi interforze che non hanno ancora terminato la loro attività. Tanto detto in linea generale, rappresento che anche la Polizia postale e delle comunicazioni è coinvolta nel riordino in questione, essendo evidente la necessità di adeguarne di adeguarne l'organizzazione alle notevoli trasformazioni registratesi nel settore. Infatti, alle tradizionali mansioni di scorta e tutela di beni e servizi postali se ne sono affiancate e sostituite altre del tutto differenti, caratterizzate da spiccate connotazioni di alta specializzazione tecnologica e orientate al contrasto del crimine informatico nelle sue forme più variegate. Muovendo da tale constatazione, il piano di razionalizzazione punta a concentrare le più spiccate e qualificate risorse professionali nei compartimenti dei capoluoghi regionali e nelle sezioni provinciali in cui operano procure distrettuali con ampia competenza in tema di reati informatici. Sottolineo, comunque, che le professionalità attualmente in servizio presso le sezioni continueranno a operare sul territorio, prevedendo tale rimodulazione un loro impiego nei reparti investigativi delle locali questure. Assicuro fin d'ora che il nuovo assetto organizzativo della Polizia postale e delle comunicazioni sarà ispirato a esclusive esigenze di efficientamento e adeguamento alla trasformazione tecnologica del Paese, senza che ne venga a soffrire la qualità del prodotto sicurezza, né la prossimità con i luoghi di residenza dei nostri cittadini. È impensabile, d'altra parte, che il Ministero dell'interno possa depauperare un servizio, quello della Polizia postale e delle comunicazioni appunto, deputato a presidiare un ambito di interesse strategico per il Paese. L'informatica e i sistemi di comunicazione sono infatti diventati strumenti di uso abituale delle associazioni criminali di tipo mafioso e terroristico e il contrasto di tali sodalizi su Internet richiede, nella logica di corrispondere simmetricamente alla minaccia, l'adeguamento costante delle tecnologie in uso, oltreché - ovviamente - dei livelli di professionalità delle risorse umane in dotazione. Infine, per quanto attiene alla chiusura della sede della Polizia ferroviaria di Modena, paventata nell'interrogazione del senatore Vaccari, informo che il progetto di razionalizzazione non prevede tale ipotesi.

rimodulazioni, previste nel piano di riordino in discussione dal 2014, prevedono la concentrazione delle competenze proprie della specialità della Polizia postale nei capoluoghi regionali e nelle sezioni provinciali ove operano procure procure distrettuali che hanno particolari competenze nel perseguire i reati informatici. Anche a nome degli altri colleghi firmatari, mi dichiaro moderatamente e parzialmente soddisfatta per la risposta ricevuta. Aggiungo che vorrei che il Ministero dell'interno tenesse ben presente la necessità di avere presidi diffusi sul territorio, proprio per agevolare le attività di indagine, permettendo una capillare conoscenza del tessuto socioeconomico locale,

furti di identità, cyberbullismo, prevenzione e indagine dei reati di pedofilia e *stalking* sono solo alcune delle attività che la Polizia postale manda avanti con accuratezza e grande dedizione, grazie alla specifica esperienza raggiunta negli anni di attività. Il *modus operandi* elaborato dalla Polizia postale rappresenta una delle buone pratiche che merita di essere valorizzata all'interno della pubblica amministrazione. Per questo motivo, si chiede di non sacrificare un'eccellenza delle Forze dell'ordine italiane, le cui capacità di indagine e prevenzione si si stanno dimostrando ai massimi livelli in questi anni in cui il terrorismo sta colpendo gravemente l'Europa, per effettuare pochi e trascurabili risparmi per le casse pubbliche, assolutamente inopportuni se si tratta di limitare la qualità dei servizi per la sicurezza dei cittadini.

Vice Ministro, la risposta è soddisfacente quanto ai chiarimenti forniti, ma c'è un problema di base. Come ha detto la senatrice Albano, i posti di Polizia postale sono quasi tutti a carico, in termini di strutture e mezzi, di Poste

un fenomeno che cresce ogni giorno e si espande a macchia d'olio sull'intero territorio della Capitanata, che è la terza Provincia d'Italia per estensione territoriale. Questo è il dato reale. Pertanto, immaginare di chiudere il presidio di Polizia postale di Foggia è qualcosa di assurdo e incredibile

Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno la senatrice Fasiolo chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'interno intenda intraprendere affinché gli uffici anagrafici dei Comuni, le Ferrovie dello Stato, l'INAIL, l'INPS, gli uffici della Motorizzazione civile e le aziende sanitarie applichino quanto previsto dalla legge n. 54 del 1989 in tema di compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace. Informo, innanzitutto, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge in questione, il Ministero dell'interno ha diramato nel tempo numerose circolari volte a sollecitare i Comuni alla sua corretta applicazione. In particolare, con la circolare n. 9 del 2005 sono state sensibilizzate tutte le pubbliche amministrazioni al rispetto dell'obbligo di riportare nei documenti rilasciati unicamente il nome italiano del Comune di nascita nonché dell'obbligo di adeguare i documenti stessi alle norme della legge anche su semplice richiesta orale del cittadino interessato. Con un'ulteriore circolare, la n. 4 del 2007, sono state coinvolte nella tematica anche le Conferenze permanenti istituite - come è noto - presso le prefetture, allo scopo di garantire il raccordo dell'attività amministrativa delle strutture periferiche dello Stato e l'attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali. Richiamo, altresì, un'altra circolare del 2007 - la n. 42 - alla quale è stato allegato l'elenco dei Comuni appartenenti ai territori ceduti e con cui sono stati invitati i prefetti a sensibilizzare «altri soggetti, quali le Ferrovie dello Stato, l'INAIL, l'INPS, gli uffici della Motorizzazione civile, le aziende sanitarie, sul corretto adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della legge». L'attenzione del Governo sul tema non è venuta mai meno, tant'è che, proprio in materia di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in territori «ceduti», il 5 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato una direttiva volta a precisare definitivamente i termini di applicazione della legge n. Evidenzio che la diramazione della direttiva è avvenuta in esito ai lavori del tavolo di coordinamento tra il Governo e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Come ricordato nell'interrogazione, tale direttiva «mira ad affermare il principio secondo cui il luogo di nascita delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento "nascita" si è verificato, Pertanto, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente hanno l'obbligo dì riportare unicamente il nome italiano del Comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene». A tal riguardo, va rilevato che, anche per ovviare a carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati che non erano in grado di riconoscere come italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto di trattati internazionali, la suddetta direttiva ha allegato «gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, nonché dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977, con la specificazione delle Province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali». La medesima direttiva ha inoltre evidenziato che, ai fini della sua applicazione, «costituisce valido strumento di ausilio il servizio *on line* di verifica del codice fiscale», disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Successivamente, con un'ulteriore circolare del 17 ottobre 2012, il Ministero dell'interno è tornato sull'argomento, ribadendo l'esigenza di assicurare la corretta applicazione della normativa in esame. Da ultimo, per completezza, informo che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è tuttora attivo un tavolo di coordinamento tra Governo e associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per l'esame congiunto di tematiche segnalate dalle associazioni medesime. Nel corso delle riunioni svolte da tale organismo, è emerso che tutti i Comuni sono allineati alle disposizioni della legge n. 54 del 1989 e che solo qualche isolata azienda sanitaria locale e qualche ufficio statale non hanno applicato le norme in questione. Nel corso dell'ultimo incontro del tavolo, tenutosi presso la Presidenza del Consiglio lo scorso 27 aprile, è stata rappresentata alle associazioni la più ampia disponibilità del Ministero dell'interno e, più in generale, del Governo a promuovere ogni ulteriore intervento per la soluzione delle problematiche ancora aperte di competenza, ivi compresi quelli utili alla positiva definizione dei singoli casi

monitorato che tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le Ferrovie dello Stato, l'INAIL, l'INPS, gli uffici della Motorizzazione civile e le aziende sanitarie, come rilevava, si attengano alle norme e agli obblighi di legge, in particolare

chiedono al Governo l'adozione di iniziative volte a mettere in sicurezza la struttura. I senatori interroganti chiedono inoltre notizie sull'eventuale trasferimento del comando a Spoltore - soluzione, questa, caldeggiata dal sindaco di quel Comune - e, più in generale, sull'individuazione di una soluzione definitiva dell'annosa questione. Le problematiche di tipo statico e igienico-sanitario relative alla sede del comando provinciale di Pescara sono ben note al Ministero dell'interno e alla Provincia di Pescara, proprietaria dell'immobile, che sono più volte intervenuti, man mano che se ne è manifestata la necessità e con oneri a carico ora dell'una ora dell'altra amministrazione, con l'effettuazione di opere di consolidamento e di manutenzione riguardanti i solai dell'edificio, le camerate, le autorimesse, a cui vanno aggiunti i lavori di rifacimento degli impianti idrici e igienici. Nel contempo, il Ministero dell'interno, tenuto conto della dichiarata impossibilità della Provincia ad affrontare le spese necessarie ad una ristrutturazione complessiva dell'immobile, ha avviato un costante confronto con le diverse amministrazioni interessate, volto a reperire un'area del capoluogo o delle zone vicine idonea alla realizzazione della nuova struttura operativa. Il confronto, a lungo infruttuoso, ha portato lo scorso anno all'individuazione di alcune possibili aree. all'Amministrazione dell'interno, la più confacente alle esigenze del comando provinciale è risultata essere quella sita nel Comune capoluogo in via Pantini, che, oltre ad essere regolare e pianeggiante, nonché priva di impedimenti, consente l'immissione rapida sia verso il territorio provinciale, tramite la circonvallazione e i raccordi autostradali, sia verso il centro cittadino. A tal riguardo, giova evidenziare che il 50 per cento degli interventi di soccorso gravanti sulla sede centrale di Pescara avviene proprio nell'area cittadina. L'area in argomento risulta essere di proprietà della RAI ed è stato attivato l'*iter* tecnico-amministrativo necessario alla sua acquisizione. è opportuno evidenziare sin d'ora - richiederà tempi non brevi. Le altre aree proposte all'Amministrazione dell'interno, tra cui quella del Comune di Spoltore, presentano una serie di inconvenienti quali: superfici irregolari, vicinanza della linea ferroviaria (circostanza che impone il rispetto di determinate distanze di sicurezza con riduzione della superficie utilizzabile), notevoli dislivelli di quota che richiederebbero opere di movimento terra e sbancamento finanziariamente onerose. Inoltre, sempre con riferimento alle predette aree, la tipologia delle strade ivi presenti e la densità di traffico durante le ore del giorno sarebbero tali da impedire ai mezzi di soccorso un rapido accesso al centro città. In particolare, l'area sita nel Comune di Spoltore, che ha il pregio di poter essere resa disponibile in tempi brevi, non è risultata idonea né dal punto di vista orografico, né, soprattutto, per la viabilità di accesso al centro cittadino. A tal proposito, si evidenzia che l'aspetto prioritario per la realizzazione della sede del comando è, oltre all'ubicazione su una superficie pianeggiante, il facile raggiungimento della stessa dagli utenti nonché l'accesso rapido al centro città, giacché il resto della Provincia è già servito da distaccamenti territoriali. Per quanto concerne, infine, la situazione di morosità nei confronti della Provincia cui si fa riferimento nell'interrogazione, informo che, a far data dal 1° gennaio 2014, l'Amministrazione dell'interno non aveva corrisposto al predetto ente quanto dovuto per la locazione. Tale situazione era stata determinata, inizialmente, dalla mancanza di fondi sul relativo capitolo per ragioni connesse alla complessiva posizione debitoria per gli immobili in locazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, successivamente, dall'intervenuta notifica, nel maggio 2015, di un atto di pignoramento presso terzi di una società creditrice dell'amministrazione provinciale. Al riguardo, si rappresenta che, in base alle disposizioni del codice di procedura civile, l'Amministrazione, quale terza pignorata, aveva l'obbligo di non disporre delle somme pignorate, che sono state quindi accantonate. Nello scorso mese di maggio, è intervenuta la definitiva estinzione del predetto procedimento esecutivo, disposta con ordinanza dell'autorità giudiziaria competente, ragion per cui il 1° giugno scorso è stato emesso l'ordine di pagamento in favore della Provincia di Pescara a sanatoria della morosità pregressa.

Prendo atto della sensibilità mostrata e ringrazio il Vice Ministro per aver predisposto quanto necessita affinché vengano scongiurati episodi pericolosi e, nel contempo, venga ridata dignità a luoghi di lavoro come la caserma Maurizio Berardinucci, destinata ad accogliere la sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pescara.

i quali chiedono di conoscere quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare affinché venga riconosciuto al personale pilota e specialista di aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del restante personale aeronavigante dello Stato. Si premette che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, dispone di personale dotato di particolari capacità tecniche e professionali, attestate dal possesso di brevetti o certificazioni rilasciate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a seguito del superamento di corsi di formazione specialistica, per svolgere le funzioni di piloti e specialisti di aereo e di elicotteri, di sommozzatori, di nautici e di addetti alle telecomunicazioni. L'esercizio di tali funzioni, fondamentali per le attività di soccorso tecnico urgente, volte a salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. In particolare, al personale aeronavigante è attualmente corrisposta un'indennità di volo, contrattualmente determinata con accordo sindacale del 22 novembre 2004, ammontante a circa 8.000 euro all'anno per i piloti e a circa 6.800 euro per gli specialisti, erogata nella stessa misura indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta o dall'anzianità di servizio. Tale indennità risulta sicuramente inferiore a quelle riconosciute all'omologo personale delle altre organizzazioni dello Stato a ordinamento militare e civile. Peraltro, l'ingresso di parte della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato e del relativo personale aeronavigante nel Dipartimento dei vigili del fuoco, a seguito dell'assorbimento disposto dalla legge n. 124 del 2015 e attuato con il decreto legislativo n. 177 del 2016, ha reso ancora più immediata ed evidente tale disparità di trattamento economico. Va fatta una breve digressione per informare che, con ulteriori provvedimenti attuativi, l'Amministrazione dell'interno, oltre a definire l'organizzazione del servizio antincendio boschivo nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco e ad articolare lo stesso servizio in strutture centrali e territoriali, territoriali, provvederà anche alla riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale. Tale riorganizzazione è indispensabile, in quanto, a seguito dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è accresciuta con il trasferimento di 96 piloti e specialisti di elicottero e 16 mezzi aerei del Corpo forestale dello Stato, che si sono andati ad aggiungere ai 19 aerei canadair acquisiti nel 2013 per effetto del passaggio dal Dipartimento della protezione civile. Per quanto ho appena detto, l'amministrazione è certamente motivata a valorizzare il personale aeronavigante del Corpo nazionale, anche sotto i profili oggetto dell'interrogazione. Ovviamente la questione non può essere affrontata senza considerare anche le altre specialità del Corpo nazionale - cioè, i sommozzatori, i nautici e i radioriparatori - il che comporterà anche un maggior impegno finanziario e la necessità di avviare un percorso per reperire le risorse necessarie allo scopo e anche per realizzare il completo allineamento agli altri Corpi dello Stato. Uno strumento utile in tal senso potrebbe rinvenirsi nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015, preordinata all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, anche attraverso il riordino degli attuali ruoli e qualifiche ruoli e qualifiche del personale. Tale delega prevede l'emanazione di un decreto legislativo e la possibilità di emanare entro un anno un secondo decreto legislativo recante disposizioni interpretative e correttive del primo. Il primo decreto legislativo - n. 97 del 29 maggio 2017 - è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno scorso ed entrerà in vigore dopodomani. Si evidenzia, al riguardo, che nella seduta del 3 maggio scorso, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in questione, tra le altre osservazioni aveva chiesto al Governo di valutare «l'opportunità di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo». Per esaminare questa osservazione e, più in generale, per approfondire tutte le questioni aperte in tema di ordinamento del personale dei Vigili del fuoco, l'Amministrazione ha già aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, nella prospettiva dell'attivazione della procedura di adozione del decreto legislativo correttivo a cui ho fatto riferimento prima. Proprio questo provvedimento correttivo appare il veicolo normativo più appropriato per affrontare la questione oggetto dell'odierna interrogazione, sostenendo il percorso di armonizzazione delle indennità di tutto il personale specialista del Corpo nazionale, compreso ovviamente quello aeronavigante.

Signor Presidente, la senatrice Nugnes, unitamente ad altri senatori, richiama l'attenzione del Governo sul maledetto fenomeno della «Balena blu», chiedendo l'adozione di iniziative volte a contrastarne la diffusione. Va subito detto che la Polizia postale e delle comunicazioni in questi ultimi mesi ha prodotto un impegno molto profondo e determinato, tanto d'iniziativa propria, quanto sulla base di specifiche segnalazioni, con iniziative tese a valutare, anche attraverso il monitoraggio della rete Internet, l'effettiva portata di questo fenomeno, che desta allarme sociale e ha avuto una vasta eco sugli organi di informazione. Tale pratica avrebbe come obiettivo, per chi la conduce in Rete in qualità di curatore, di coinvolgere i partecipanti in atti di autolesionismo, inducendo comportamenti sempre più pericolosi fino a determinare nelle vittime intenzioni suicide. L'attività della Polizia postale e delle comunicazioni mira ad identificare persone o gruppi di persone eventualmente coinvolti in tale fenomeno, per prevenire l'esposizione di bambini e ragazzi ad un rischio per la loro incolumità connesso alla frequentazione della Rete. Nel contempo, ai medesimi fini, viene svolta una raccolta centralizzata delle segnalazioni. La Polizia postale e delle comunicazioni ha ricevuto finora circa 170 segnalazioni relative al fenomeno. Gli accertamenti disposti, volti alla tempestiva localizzazione delle vittime, hanno fatto emergere che la percentuale dei casi qualificanti ipotesi di reato, come l'istigazione al suicidio o il procurato allarme, è inferiore al 5 per cento delle segnalazioni pervenute. Informo che nel portale del commissariato di pubblica sicurezza *on line* è stata resa operativa una stanza virtuale dedicata, per rivolgere consigli ai genitori e ai ragazzi e illustrare i pericoli emergenti in Rete, Rete, agevolare le segnalazioni e sensibilizzare gli utenti, anche grazie all'ausilio specialistico di psicologi della Polizia di Stato. È peraltro evidente che la prevenzione di qualsiasi forma di uso distorto o pericoloso del *web* che costituisca espressione di disagio e vulnerabilità giovanile compreso il fenomeno qui in esame - richiede anche il coinvolgimento attivo del mondo della scuola, delle famiglie e dell'associazionismo. In tal senso, la tematica della «Balena blu» è stata inserita nella campagna che gli uffici della citata struttura specialistica della Polizia di Stato svolgono nelle scuole per un uso consapevole del *web*. Assicuro che la Polizia postale continuerà a monitorare assiduamente la rete Internet per prevenire e contrastare la diffusione di tale fenomeno, riferendo prontamente all'autorità giudiziaria sui contenuti di rilevanza penale eventualmente rinvenuti all'interno degli spazi e servizi di comunicazione *on line*. Quanto all'episodio menzionato nell'interrogazione, relativo al suicidio di un quindicenne, avvenuto nella città di Livorno nello scorso mese di febbraio, confermo che gli accertamenti svolti dalle forze di polizia, supportati anche da numerose informazioni testimoniali, hanno condotto ad escludere l'ipotesi, sostenuta da alcuni *media*, che l'evento fosse riconducibile al fenomeno in questione. Il pubblico ministero titolare del fascicolo sull'evento, all'esito delle indagini, ha chiesto ed ottenuto l'archiviazione del relativo procedimento.

l'accertamento della sussistenza del fenomeno nello specifico. Lei ha parlato di 170 170 segnalazioni e di un 5 per cento di tali segnalazioni che si sono poi tramutate in ipotesi di reato, ma non ha detto se il fenomeno sia riconducibile effettivamente all'ipotesi di questo programma specifico che coinvolgerebbe i ragazzi. Sono sicuramente confortata dal fatto che la Polizia postale stia indagando e di poter dare risposta a chi ci sollecitava in tal senso.

infatti, deve essere fatto nei luoghi da loro frequentati e tramite gli strumenti loro più consoni, con il supporto psicologico che è sia per l'uso della rete, che per per quanti altri problemi possano interessare gli adolescenti, in questa fase così complicata del loro passaggio all'età adulta. all'età adulta. Sono sufficientemente soddisfatta anche se, chiaramente, un accertamento di una negazione del fenomeno mi avrebbe maggiormente tranquillizzato, ma purtroppo non è così.